che coinvolgono il MAECI nel raggiungimento dei previsti saldi di finanza pubblica e nella riduzione del debito e impongono necessariamente una revisione della politica sugli immobili demaniali. Dapprima, la legge di stabilità del 2016 ha stabilito che il MAECI versi all'entrata del bilancio dello Stato 20 milioni di euro per il 2016 e 10 per il 2017 e il 2018 tramite operazioni di dismissioni immobiliari di beni non più utili per le finalità istituzionali. Successivamente, la legge di bilancio 2017 ha incrementato tali cifre, stabilendo che il MAECI dovrà conseguire dalle dismissioni immobiliari proventi per 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mentre per il 2019 è stato inserito un *target* di 16 milioni di euro. Con le medesime disposizioni, la legge ha altresì previsto che, in caso di mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi, siano decurtati i fondi per un ammontare corrispondente destinati all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo. Poiché a nessuno sfugge l'importanza che l'attività di cooperazione ha per la politica di questo Ministero, si comprende come la dismissione del patrimonio immobiliare abbia conseguenze ben più ampie di quanto si possa immaginare. Venendo alla situazione particolare a Monaco di Baviera, tengo innanzi tutto a sottolineare - e vorrei che fosse chiaro - come non sia mai stata presa in considerazione una limitazione delle attività del consolato generale né tanto meno una sua chiusura. Non sarebbe del resto possibile in considerazione della grande collettività italiana ivi residente e dell'importanza della città di Monaco di Baviera e del Land, la Baviera in generale, non solo nel contesto tedesco, ma anche in ambito europeo. Altra cosa è lo stabile che ospita il consolato generale: occorre prendere atto che non è totalmente funzionale alle attività istituzionali, a causa delle sue condizioni e della necessità di interventi strutturali. è stata esplorata la possibilità, con avviso pubblico, di permuta con conguaglio, ma la procedura è stata temporaneamente accantonata, non avendo prodotto i risultati sperati. Si continua tuttavia a ritenere che sia nell'interesse pubblico procedere all'alienazione dell'immobile, tenuto conto del valore di mercato dello stabile e delle necessità istituzionali. Vorrei rassicurare sul fatto che un'eventuale vendita sarà comunque subordinata alla preventiva individuazione di locali idonei, altrettanto o più funzionali, dove ricollocare le strutture. Nella scelta del nuovo edificio si terrà inoltre conto di aspetti importanti come la centralità della sede, la sua accessibilità al pubblico, le garanzie di sicurezza sul lavoro e gli *standard* di efficienza energetica. Quanto alla convenienza dell'operazione immobiliare, per la perizia dell'immobile si è provveduto secondo quanto previsto dalla legge n. 183 del 2011, avvalendosi di *expertise* locale in condizioni di indipendenza e assenza di interesse.

La procedura per manifestazione di interesse ha avuto esito negativo. È stato, quindi, indicato alla sede di dare la massima pubblicità alla vendita per poi procedere a trattativa privata. Da allora risultano pervenute e sono state esaminate dalla sede alcune offerte di acquisto presentate da potenziali acquirenti in linea con il parametro indicato dalla stima di valore aggiornata al 2016, dell'importo di 2.150.000 euro. Sono in corso gli accertamenti di rito giuridici e finanziari per verificare la capacità dei potenziali acquirenti a contrarre senza impedimenti. con la predisposizione di una bozza di atto di compravendita da sottoporre alla verifica finale dell'Amministrazione, non appena completati gli adempimenti necessari. Concludo dicendo che la notizia di una possibile vendita dell'edificio che ospita l'Istituto italiano di cultura di Monaco di Baviera è infondata. Non vi è alcuna istruzione della Farnesina in tal senso, tanto più che la manifestazione di interesse

Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Della Vedova per la relazione su un tema che raramente è oggetto di confronto parlamentare, malgrado il numero di atti presentati sia da me che dal senatore Micheloni. Potremmo definirlo proprio il «paradosso di Monaco», vale a dire la scelta di dismettere le strutture di rappresentanza, rimodulandone le potenzialità in un momento storico-sociale in cui la domanda di servizi cresce in maniera esponenziale, anche in virtù - lei l'ha segnalato molto bene - degli esiti della Brexit. Sarebbe, però, opportuno porre l'accento sulle altre criticità funzionali del consolato di Monaco che facevano parte della mia ben più articolata La chiusura nel 2014 dello sportello di Norimberga, che serviva circa 32.000 connazionali, ha condotto all'assorbimento del bacino di utenza da parte di Monaco, presso la cui struttura però è stata anche operata una riduzione del personale. elementi sono stati segnalati più volte nel corso degli anni, tanto da condurre il sottoscritto insieme ad altri, come il collega Micheloni, a suggerire l'individuazione di un interlocutore consolare nelle città satelliti di Monaco, *in primis* Norimberga, dove tra l'altro esiste una struttura a uso gratuito per eventuali installazioni, al fine di alleggerire la mole di lavoro di Monaco e agevolare le migliaia di cittadini che da Norimberga e zone limitrofe sono costretti a dirigersi a Monaco, percorrendo anche 300 chilometri, per un semplice rinnovo di passaporto. Anche perché risulta che al momento sia di circa sei mesi il tempo di attesa per un rinnovo passaporto. Certamente, leggendo gli annuari statistici della Farnesina emerge una riduzione dei servizi resi dal consolato, quasi si trattasse di una domanda che si riduce. Si omette, invece, che il ridimensionamento è correlato alla riduzione di unità che, ridotto, opera sicuramente in misura minore. Perciò vincolare le ragioni della razionalizzazione a quelle del ridotto numero di servizi consolari appare come un falso amministrativo. Il fatto stesso che sui territori oggetto di razionalizzazione consolare vengano poi favorite altre forme di rappresentanza, come consolati onorari e patronati, evidenzia come l'amministrazione sia consapevole del vuoto che le chiusure consolari stanno determinando. Il lavoro svolto dai patronati merita certamente rispetto e attenzione quale consolidata interfaccia tra cittadini oltre confine e istituzioni in sede, come l'INPS. Ma è cosa ben diversa da quello a cui stiamo assistendo oggi, vale a dire la tendenza a demandare al patronato attività finora di esclusiva competenza delle autorità diplomatiche e consolari, come la gestione del rilascio dei passaporti. Questa crescita esponenziale di patronati nei territori stranieri sembra ratificare una delegittimazione del ruolo di garanzia svolto dallo Stato in ambiti delicati come l'assistenza ai nostri connazionali, attraverso l'attivazione di una delega - dalla opaca legittimità normativa - in capo ad un soggetto privato, nel momento esatto in cui lo Stato stesso ritiene di non poter avere gli strumenti per portare avanti quel ruolo. Una struttura privata non può e non deve essere una diretta emanazione dello Stato italiano, in totale deroga rispetto a quanto sancito dalla norma, poiché comporterebbe una violazione dei dettami di garanzia e trasparenza che soltanto l'istituzione nazionale può garantire. Un'ulteriore riflessione va fatta in riferimento al ruolo del console onorario, il quale però, in ragione del carattere volontario dell'incarico e delle limitazioni di carattere normativo, non può sostituirsi un servizio consolare, soprattutto quando il bacino di utenza è tanto vasto. Ricordo che il numero dei nostri connazionali che si presentano mediamente al ricevimento del consolato onorario si attesta sulle 40 unità nel periodo invernale, per raggiungere le 80 unità nella stagione estiva. Parliamo dunque di un carico di lavoro che non può essere sostenuto su base volontaria e non si può lasciare nelle mani di un profilo che non ne detiene la legittimità e le competenze adeguate. Inoltre, l'amministrazione ha più volte fornito rassicurazioni circa la volontà di garantire la permanenza della struttura consolare nell'attuale immobile, ma di contro le voci voci di continue perizie di valore nel corso degli ultimi tre anni, unitamente alle voci di una decisione di trovare un immobile più piccolo, sono elemento di insicurezza per i connazionali. Signor Sottosegretario, malgrado le evidenze da lei segnalate, si fatica a capire la traccia dell'analisi costi-benefici sottesa a tali progetti, e se ve ne sia qualcuna alla base delle operazioni di razionalizzazione attuate al momento in Germania. L'ultimo capitolo va rintracciato nella sospensione dell'esperimento del funzionario itinerante a Norimberga, riconducibile, tra le altre cose, alla limitata disponibilità di personale da dirigere in sede da parte della struttura di Monaco, già in evidente sofferenza. Tutto questo per dire che i parametri e i calcoli che noi abbiamo effettuato con le comunità e gli organismi di rappresentanza propendono per un'assoluta antieconomicità di una dismissione immobiliare, non presa come una operazione a sé stante, ma estrapolata dal descritto scenario, in quanto atto conclusivo di un progetto poco funzionale. Su questo si auspica un confronto ampio e costante con le comunità locali, per individuare soluzioni effettivamente orientate alla tutela della corretta erogazione dei servizi consolari, al momento fortemente compromessa. L'invito al dialogo e al mutuo confronto rappresenta la priorità. Sono certo che lei, signor Sottosegretario, con la sua sensibilità potrà dare un valido contributo.

Signor Presidente, con riferimento all'atto parlamentare dei senatori Battista e altri, inerente alla vicenda del signor Colautti, dipendente della società Wärtsilä SpA, si rappresenta quanto segue. Dalle informazioni acquisite presso il competente ufficio dell'Ispettorato nazionale del lavoro risulta che il signor Colautti è stato assunto nel 2005 dalla Wärtsilä SpA in qualità di addetto alle lavorazioni meccaniche con un contratto di inserimento successivamente trasformato in contratto a tempo indeterminato. Dopo aver ricoperto l'incarico di segretario provinciale della FIOM, con conseguente aspettativa sindacale, il signor Colautti ha aderito, negli ultimi due anni, alla organizzazione USB, usufruendo di un ulteriore periodo di aspettativa. Il 6 giugno 2017, al termine del periodo di distacco, la società ha disposto il trasferimento del lavoratore dalla sede originaria di Trieste a quella di Taranto. Per quanto riguarda le motivazioni del trasferimento, i vertici aziendali hanno comunicato che nella sede di Trieste non esiste più il reparto di montaggio e assemblaggio al quale il lavoratore era stato originariamente assegnato. A Trieste, infatti, vi sono soltanto la sede legale della società e un magazzino, mentre l'attività di montaggio e assemblaggio viene svolta nella sede di Taranto (ove peraltro è in corso una commessa con la Marina militare). L'organizzazione sindacale cui appartiene il lavoratore lamenta, invece, che il trasferimento configuri una condotta antisindacale. Ciò posto, il Ministero della giustizia - espressamente interpellato dal Ministero del lavoro che rappresento - ha riferito che, lo scorso 3 luglio, il signor Colautti ha presentato, presso il tribunale di Trieste, ricorso ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile nei confronti della società Wärtsilä SpA. Con l'atto introduttivo, il ricorrente ha chiesto la declaratoria di illegittimità del proprio trasferimento dalla sede di Trieste a quella di Taranto, in quanto discriminatorio o ritorsivo o, comunque, per per inesistenza di effettive e reali ragioni tecniche e produttive, ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Lo scorso 28 luglio si è tenuta la prima udienza del procedimento cautelare, all'esito della quale il giudice su istanza congiunta delle parti - ha fissato, lo scorso 11 settembre, una seconda udienza finalizzata all'esperimento di un tentativo di conciliazione. L'udienza è stata successivamente rinviata, per i medesimi incombenti, al prossimo 25 settembre. Pertanto, in caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, ogni valutazione in ordine alla legittimità del comportamento posto in essere da Wärtsilä SpA sarà rimessa alle statuizioni definitive della competente autorità giudiziaria.

Sono un po' perplesso in merito alla motivazione data dall'azienda che sembra definire la sede di Trieste come un mero magazzino quando non lo è.

da parte del Governo che della Regione. Esiste infatti un progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentato dalla società Wärtsilä

in una sede molto lontana. È ovvio che questo sia un atto discriminatorio e non può neanche valere che questa sia una ritorsione, perché lo stesso signor Colautti ha svolto l'incarico di delegato di fabbrica per nove anni e si è reso parte

Signor Presidente, rispondo al quesito posto nell'atto in discussione fornendo i seguenti elementi. Il richiamato regolamento che, in attuazione della riforma introdotta con la legge di stabilità 2016, disciplinerà

in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 24 marzo scorso. In data 3 luglio, il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sullo schema di recante il citato regolamento, il quale è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri nella seduta del 7 agosto scorso.

Vorrei sottolineare che i ritardi a cui si fa riferimento nell'atto degli interroganti saranno in gran parte recuperati grazie alla nuova procedura prevista per il bando, che sarà totalmente *on line*, riducendo i tempi di esame e istruttoria delle relative richieste. Inoltre, giova sottolineare che, nelle more dell'approvazione, il Governo ha aumentato le risorse complessivamente a disposizione delle emittenti locali, che, a legislazione vigente, per il 2016 sono state pari a 40.800.000 euro. A queste si sono aggiunti i fondi della quota di extra gettito del canone di abbonamento RAI previsti dalla legge di stabilità 2016, in un'azione di rafforzamento delle politiche di sostegno e di qualificazione dell'emittenza radiotelevisiva, riformando così una disciplina dei contributi risalente al 2002, ormai obsoleta e inadeguata. Riguardo ai contributi relativi all'anno 2015, le procedure di liquidazione dei medesimi alle 456 emittenti televisive, risultate beneficiarie sulla base delle graduatorie approvate dai Corecom regionali, sono state avviate nello scorso mese di aprile dal Ministero e sono in fase di avanzato svolgimento. Sul sito del Ministero, nella sezione dedicata alla trasparenza, è pubblicato l'elenco delle 300 emittenti televisive cui sono già stati assegnati i contributi e i relativi importi. Queste informazioni vengono aggiornate dal Ministero con cadenza mensile. Tale attività ha avuto luogo subito dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di riparto tra le Regioni dello stanziamento complessivo di competenza per Queste procedure sono state le ultime regolate dalla vecchia normativa. Come è stato riferito in Commissione lo scorso febbraio, il ritardo per l'entrata in vigore dei decreti di riparto a livello regionale dello stanziamento non è ovviamente da imputare al Ministero ed è il motivo principale Di certo, il meccanismo complesso delle graduatorie regionali rappresenta un passaggio che ha generato anche in passato ritardi, derivanti da contenziosi ai TAR sulle singole graduatorie regionali, bloccando per mesi il processo complessivo. Con il nuovo regolamento si avvia un percorso virtuoso, che consentirà di rafforzare il sostegno al settore delle emittenti locali, in un'ottica di stimolo delle attività di editoria e di informazione, grazie a nuovi meccanismi e criteri di selezione che premiano i soggetti che investono nell'attività editoriale di maggiore qualità. La legge di stabilità 2016 ha infatti stabilito che i quattro principi in base ai quali sono definiti i criteri di erogazione sono la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno all'occupazione del settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti, l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative. La previsione che il Ministero fa con l'applicazione del nuovo regolamento è che nell'arco temporale di non più di cinque o sei mesi vengano pubblicati i bandi di gara per le annualità 2016, 2017 e 2018.

quindi una funzione decisamente fondamentale e di conseguenza la possibilità di avere delle risorse diventa vitale.

dati e argomenti che il MISE ha già fornito in sedi istituzionali diverse e che dunque immagino siano già noti. Wind Tre, azienda nata a seguito di un processo di fusione che ha interessato Wind Telecomunicazioni SpA e H3G SpA, costituisce il primo operatore nel mercato mobile in Italia,

Dalla fusione delle due società sono scaturite delle fisiologiche sovrapposizioni strutturali anche in termini di risorse. Successivamente alla fusione, Wind Tre ha gestito il processo di integrazione degli organici esclusivamente su base volontaria, utilizzando risorse proprie con le quali sono stati incentivati dipendenti che hanno manifestato interesse. L'operazione di cessione del ramo si inquadra dunque in questo ambito. Il ramo d'azienda svolge servizi di assistenza amministrativo-commerciale e tecnica di primo livello (principalmente informazioni sulla copertura della rete di telecomunicazioni). Wind Tre ha precisato di aver compiuto un'attenta verifica dei soggetti imprenditoriali che operano nel settore al fine di ricercare una controparte qualificata, finanziariamente solida, dotata di comprovata e pluriennale esperienza nel settore e di idonea struttura imprenditoriale, alla quale poter affidare lo svolgimento del servizio di *call center*. La scelta della società è caduta su Comdata, azienda da anni attiva nei settori della progettazione e gestione in *outsourcing* di sistemi e servizi. - secondo quanto evidenziato da Wind Tre - tra le aziende più stabili del settore sotto il profilo finanziario ed è in via di espansione anche oltre i confini nazionali. L'azienda ha nel proprio organico 36.000 dipendenti (di cui 6.514 in Italia al 30 aprile 2017, organico cresciuto nel 2015 e nel 2016 di un più 7,3

Il 22 maggio scorso, a seguito delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali, Wind Tre ha presentato il proprio *business plan* e in tale circostanza - come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore delle telecomunicazioni - ha anticipato l'intenzione di procedere alla cessione di ramo d'azienda, avendo come oggetto il *call center* 133 per la clientela *consumer* del *brand* Tre, illustrandone le motivazioni. Il 9 giugno 2017 Wind Tre, insieme a Comdata, ha attivato la procedura di consultazione sindacale prevista dalla normativa di legge finalizzata all'individuazione di soluzioni atte a fornire ogni più opportuna garanzia occupazionale. L'obiettivo, contestualmente alla cessione del predetto ramo d'azienda, era quello di sottoscrivere un contratto con durata settennale di fornitura da parte di Comdata di servizi di *call center*, per lo svolgimento dei quali la predetta società si sarebbe avvalsa del ramo d'azienda acquisito. Questa decisione avrebbe comportato un consolidamento dei rapporti commerciali già esistenti tra le due società e determinato un significativo rafforzamento della posizione di Comdata nel mercato dei *contact center* in Italia. Con specifico riferimento a quanto detto in premessa, in particolare alla preoccupazione espressa dagli interroganti circa il mantenimento delle garanzie occupazionali e contrattuali faccio presente che in data 27 giugno 2017 Wind Tre, Comdata e le rappresentanze sindacali unitarie di Genova, Cagliari Roma e Palermo, assistite da CGIL, CISL e UIL nazionali e territoriali, unitamente al coordinamento nazionale delle rappresentanze sindacali unitarie di Wind Tre, hanno sottoscritto un verbale di accordo con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2112 del codice civile, si è previsto il trasferimento a Comdata dei dipendenti Wind Tre occupati nel ramo d'azienda a far data dal 5 luglio 2017. Tutti i lavoratori sono stati trasferiti a Comdata senza soluzione di continuità e con mantenimento dell'anzianità di servizio, del livello di inquadramento e della pausa retribuita per la refezione nell'ambito delle otto ore per il personale *full-time* turnista. Comdata garantirà la stabilità occupazionale per tutta la durata del contratto di appalto di servizi di durata settennale con riferimento ai lavoratori che, *ex* articolo 2112 del codice civile, passeranno alle sue dipendenze per effetto della cessione di ramo d'azienda, oltre ad assicurare il mantenimento dell'attuale sede di lavoro dei lavoratori trasferiti di Cagliari, Genova, Palermo e Roma per tutta la durata del predetto contratto. Comdata, in considerazione dello sviluppo previsto del *business*, si è poi impegnata ad accogliere le richieste di incremento fino a sei ore giornaliere da parte dei *part-time* attualmente in servizio con contratti a quattro o cinque ore L'accordo prevede anche che, in caso di cessazione anticipata del contratto, Wind Tre applicherà la clausola sociale di garanzia in favore di questi lavoratori, impegnandosi a individuare un nuovo operatore che garantisca la salvaguardia dei posti di lavoro secondo quanto disposto dalla contrattazione nazionale di categoria, nell'ottica di perseguire il mantenimento dei livelli occupazionali e di trattamento. I lavoratori interessati dal trasferimento del ramo d'azienda manterranno inoltre l'iscrizione al fondo di previdenza complementare, secondo le modalità e le condizioni previste del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro delle telecomunicazioni, e rivestiranno la qualifica di socio beneficiario del fondo di solidarietà Wind Tre per tutta la durata del contratto di appalto di servizi. Per l'anno 2017, gli stessi lavoratori potranno beneficiare del pagamento del premio di risultato di Wind Tre qualora i risultati consuntivati consentano di procedere alla sua erogazione. L'accordo prevede, altresì, che agli stessi lavoratori Comdata riconosca tre giorni di permesso retribuito su base annua per malattia del bambino fino agli otto anni di età e che fino al trentaseiesimo mese di vita del bambino le mamme lavoratrici non prestino servizio di sabato. In considerazione di quanto appena riferito, emerge che i termini dell'accordo hanno, quindi, posto un'attenzione importante agli aspetti occupazionali e contrattuali relativi ai lavoratori coinvolti nella cessione del ramo d'azienda. In conclusione, vorrei assicurare che, per gli aspetti di propria competenza, il Governo e, in particolare, il Ministero dello sviluppo economico, pur rispettando evidentemente l'autonomia delle parti, continuerà a monitorare il processo di contrattazione e gli sviluppi di questa importante operazione nel settore dei *call center*.

pronunciamento sulla compatibilità di quelle esternalizzazioni annunciate il 22 maggio da parte della neocostituita società Wind con gli obiettivi di tutela del futuro occupazionale dei lavoratori impiegati nel servizio clienti. Devo riconoscere che in questa vicenda il Governo ha avuto un ruolo determinante nella difesa di quei posti di lavoro e, in particolare, dei lavoratori di quei siti che sono stati ricordati (Genova, Cagliari, Roma e Palermo), che sarebbero stati coinvolti in un percorso di cessione di ramo d'azienda - diciamoci la verità

persuasivo che il Governo ha fatto. Bene fa il Governo a monitorare nei prossimi mesi anche la situazione la situazione dell'applicazione di quell'accordo. Noi ci permetteremo di continuare, come parlamentari, sorvegliare lo stato dell'applicazione dell'accordo tra lavoratori e azienda e, in particolare, di quella parte che garantisce il posto ai lavoratori lavoratori coinvolti per tutta la durata del contratto di fornitura di servizi garantito da Wind a Comdata, che ha una durata di sette anni. E noi saremo molto molto attenti che quell'accordo venga completamente portato avanti fino alla conclusione del contratto stesso. Ovviamente ci auguriamo, per le prospettive della telefonia del nostro Paese, in quanto stiamo parlando del più grande gruppo del settore del nostro Paese, e per le prospettive di lavoro dei lavoratori coinvolti, che si vada anche oltre il settennio.